la nostra dichiarazione di voto, anche se probabilmente andrò oltre il minuto che avevo chiesto ieri sera per fare la stessa cosa.

all'istituzione di un'autorità di controllo e certificazione dei bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni

quasi fosse un confronto interpersonale, a volte ristretto addirittura al collega Morando e al sottoscritto. In realtà, è un argomento portante della democrazia, e della democrazia economica: chiediamo alle aziende di certificare i bilanci,

Grazie

aprì un dibattito molto serio sull'argomento. A pochi passi da quest'Aula, a piazza Sant'Andrea della Valle, nell'ambito di un'istituzione privata (un centro studi chiamato AREL,

rappresentanti delle istituzioni di altri Paesi furono presenti al dibattito e dettero contributi di esperienza: tra questi il direttore generale del CBO *(Congressional Budget Office)*, struttura che svolge questo ruolo incastonata all'interno del Congresso americano, così come il collega Morando ha ricordato ieri.

ma che l'argomento sarebbe stato affrontato con maggiore approfondimento in tempi successivi, e così tale previsione

Ovviamente, è la sostanza che conta, cioè la certificazione dei bilanci pubblici, che è il motivo per il quale noi ieri abbiamo votato a favore dell'emendamento illustrato dal collega Morando.

il debito pubblico italiano è esploso, ma forse non tutti hanno avvertenza che un terzo del debito pubblico italiano, cioè oltre 600 miliardi di euro di quel debito che ci troviamo oggi

Ed è semplice fare questo calcolo: basta vedere, nell'arco di questi 35 anni, le cosiddette operazioni di debiti pregressi. Il trucco è consistito nel non far emergere i debiti nel bilancio dell'anno, accumularli nascosti per qualche anno, e ogni quattro, cinque anni, di fronte all'evidenza, farli emergere come debiti pregressi, con la tecnicalità truffaldina di metterli - come si dice - sotto la linea. Cari colleghi, metterli sotto la linea significa farli emergere senza passare in un bilancio. Questa tecnica truffaldina

correttamente informato da un'*authority* interna o esterna ad esso, almeno se ne avrebbe avuta consapevolezza.

Senza quei trucchi avremmo avuto, come Parlamento, in questi 35 anni, la consapevolezza, e la possibilità, con chiarezza e trasparenza e certificazione dei dati, di avere l'evoluzione del debito pubblico tedesco. Come vede, signor Presidente, cari colleghi, non è una questione interpersonale ridotta al dibattito fra il collega Morando, il sottoscritto e pochi altri addetti: è un tema centrale della politica, e della politica economica. Purtroppo, come ho già ricordato ieri, abbiamo non solo questo enorme arco di tempo di 35 anni, ma anche esempi concreti clamorosi e recenti, che riguardano ogni tipo di coalizione di Governo. Citerò due esempi: il primo riguarda il Governo di centrosinistra Prodi, quando in quest'Aula venne il sottosegretario Sartor con una lettera a sua firma che pretendeva di sostituire la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato su un provvedimento. Sempre in queste Aule, nelle settimane scorse abbiamo visto certificazioni relative a provvedimenti - mi riferisco alla cedolare secca sugli affitti palesemente scoperti ma coperti con una foglia di fico, cioè la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, dipendente dal Ministero dell'economia, che improvvisamente,

aritmeticamente determina in quello stesso anno una perdita di gettito che la Ragioneria aveva stimato in precedenza in 2,8 miliardi di reddito

trasforma la perdita di gettito che aritmeticamente c'è (anche se è ovvio che poi l'emersione degli affitti determinerà maggiore gettito), e quei meno 2,8 miliardi di perdita di gettito sono trasformati in più 3 miliardi di maggior gettito, proveniente dall'emersione degli affitti, già nell'anno di grazia 2011, cioè quest'anno, e siamo ad aprile! questi due esempi dimostrano che, senza la certificazione dei bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni, non solo il Parlamento decide senza avere la corretta informazione, ma viene meno il pilastro della democrazia politica ed economica,

del CBO americano che aveva suggerito il senatore Morando, sia nella formulazione che discutiamo adesso dell'autorità indipendente, significa assumere la responsabilità di proiettare nei prossimi anni le stesse identiche condizioni degli ultimi trent'anni che hanno determinato le condizioni del debito pubblico. Allora, chi pontifica sulla gravità del debito pubblico lo fa a ragione, chi pontifica sulla necessità degli equilibri finanziari lo fa a ragione: queste persone si assumano la responsabilità di di poggiare la prima pietra fondante, che è l'autorità di controllo. Se dicono "no", se il Governo dice "no" a questo, allora è vano assumere la facciata del rigore dei conti pubblici: quella è solo un'etichetta per nascondere i giochi delle tre carte che vengono fatti all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, qualunque sia il Governo del momento,

controllare le politiche fiscali ed io credo che questa potrebbe essere davvero la svolta che attendiamo, se avremo il coraggio di votare favorevolmente a questo emendamento, come peraltro anche a quello presentato dai senatori Lusi e Morando nel pomeriggio di ieri.

Signor Presidente, nel giugno 2009, quando è stata votata la legge n. 196 di cui oggi stiamo discutendo le modifiche, il Gruppo dell'Italia dei Valori espresse il proprio voto favorevole sulla riforma della legge di contabilità. Lo facemmo però senza alcuna enfasi o retorica, perché per noi non era una priorità del Paese, anche se era comunque una necessità: una necessità se veniva subordinata al quadro degli obblighi comunitari di cui abbiamo parlato ampiamente nel corso della discussione, e più in prospettiva del federalismo fiscale. un aspetto politico centrale di tutta la nostra proposta è stato il rapporto tra Governo e Parlamento, ossia porre rimedio nelle procedure finanziarie e nelle regole contabili allo squilibrio tra una adeguata responsabilità del Governo, che pure deve esserci, e gli strumenti di controllo, di indirizzo e di decisione che devono essere messi a disposizione del Parlamento.

Si è sentita la necessità dell'intervento autorevole del presidente della Repubblica Napolitano, che, in occasione del decreto milleproroghe, ha paventato quella che lui stesso ha definito, con parole preoccupanti, una compressione del ruolo del Parlamento.

da questo Governo per nascondere una maggioranza sempre più confusa e divisa sulle cose da fare, ottenendo l'effetto di marginalizzare sempre di più il ruolo del Parlamento nelle decisioni di finanza pubblica.

ce ne hanno parlato poco fa anche alcuni colleghi intervenuti - di tutti i processi che concorrono al miglioramento della conoscenza, della trasparenza, del monitoraggio e del controllo dei conti pubblici. qui sappiamo come è andata a finire, e a distanza di oltre un anno il presidente dalla Corte dei conti Giampaolino lo ha ribadito proprio in questi giorni. La Corte La Corte continua ripetutamente a sottolineare, nelle relazioni quadrimestrali sulla legislazione di spesa, le carenze informative delle relazioni tecniche, e in particolare quelle legate ai provvedimenti legislativi d'urgenza, troppo spesso sono prive dei necessari chiarimenti che servono al Parlamento. Poi, il risultato è davanti agli occhi di tutti: nel corso degli anni, come ha ricordato poc'anzi il senatore Baldassarri, è stata pressoché impossibile

di poter mettere un freno alla spesa con strumenti di intervento di contenimento automatico, i cosiddetti, famigerati tagli lineari, che, senza distinguere ciò che favorisce la crescita e ciò che la ostacola (senza alcuna distinzione tra chi deve dare di più e chi invece deve essere sostenuto), hanno finito per penalizzare i settori vitali del nostro Paese, determinando per giunta, secondo l'ISTAT, un ulteriore aumento della spesa pubblica. Vede, Presidente, questa per noi era una premessa necessaria per spiegare le ragioni che all'epoca ci hanno indotto a votare a favore della legge n. 196 del 2009, così come

devono concorrere al coordinamento delle politiche di bilancio dei Paesi dell'Unione europea. Ciò deve avvenire prevalentemente su due aspetti: la tempistica di presentazione, ragion per cui ci adeguiamo alla famosa sessione europea di bilancio, e il contenuto di alcuni importanti documenti finanziari. Il nostro voto sarà favorevole, però lo dichiaro con la stessa disillusione di allora, nonché con una preoccupazione ancora più grave, oggi. Noi sappiamo bene - i precedenti che ho ricordato poc'anzi lo dimostrano - che il rafforzamento delle regole, quantunque necessarie e vincolanti, non è di per sé una misura sufficiente, e la loro reale efficacia dipenderà dalla capacità di ogni Paese di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. Ebbene, il problema è proprio questo: la manifesta irresponsabilità dell'attuale Governo del nostro Paese. Negli ultimi due vertici europei, che faranno da piattaforma per il prossimo incontro che si terrà il 25 marzo, sono state prospettate soluzioni che per noi costituiscono un importante punto di partenza, su cui dovremo riflettere e ragionare un po' tutti. Cosa ci chiede l'Europa? Un impegno di notevole rilievo politico. Tenere in ordine i conti dello Stato è importante,

ha la responsabilità di governo ha anche il dovere di spiegare al Paese le sue scelte. Allora, il dato politico nuovo che cogliamo è che il Patto per l'euro il Patto per l'euro va al di là dei soli criteri sui saldi di finanza pubblica: abbiamo parlato di *deficit* al 3 per cento, di debito al 60 per cento, ma il Patto per l'euro ha il merito di porre all'attenzione dei Governi i problemi strutturali delle economie

europeo, in aggiunta a quanto detto ampiamente in discussione, delinea molte aree di intervento e contiene numerose indicazioni importanti, sul mercato del lavoro, sul sistema previdenziale, sul controllo dei costi del settore pubblico; ma ancora più rilevante è il fatto che l'Europa stessa ci dia indicazioni chiare sugli investimenti nella scuola, nella ricerca e nella formazione, cioè proprio quei settori che sono stati oggetto di attenzione da parte del Governo in ben altra direzione. Abbiamo davanti tempi molto ristretti: una delle prime scadenze sarà il 10 aprile, con la presentazione in Parlamento del Documento di economia e finanza. La stessa scadenza per l'aggiornamento del Programma, che non a caso si chiama di stabilità e di crescita, non solo con gli obiettivi di finanza pubblica che sono stati ricordati, ma anche con i principali indicatori che sono alla base delle decisioni di politica economica che dovranno essere adottate. Infine, nel testo dovrà essere inserito lo schema del Programma nazionale di riforma che, al pari di ogni altro Paese, dovremo inviare a Bruxelles in versione integrale entro fine aprile,

Ci avviciniamo a questa scadenza con un debito pubblico che continua a macinare record: ogni famiglia ha sulle spalle 90.000 euro di debito. Gli italiani versano più tasse rispetto a quanto ricevono in termini di servizi, e lo faranno ancora di più con il federalismo truccato truccato che abbiamo approvato tempo fa. I nostri disoccupati sono i meno aiutati d'Europa e i salari d'ingresso dei giovani sono fermi da oltre dieci anni, con un tasso di disoccupazione giovanile che tocca il 30 per cento: questo è il quadro

il Ministro dell'economia, che invece continua a parlarci, dopo 16 anni, di una rivoluzione liberale di cui non c'è traccia e che lui stesso non sa in cosa consista.

è completamente assente sulle politiche economiche europee, compreso il Presidente del Consiglio, che dovrebbe lavorare più di giorno che di notte.

economica, che consiste nel cambiamento di una trentina di parole della Costituzione, in un'insalata russa di provvedimenti marginali, quasi tutti di spesa: dall'eterna banda larga, sempre presente, al piano casa, che viene ripreso e ripescato, cercando di far credere che tutto questo possa aumentare

una buona azione riformatrice richiede due condizioni: la prima è sapere quello che si vuole fare; la seconda è che si utilizzino i mezzi e gli strumenti adeguati per poterlo fare.

voteremo a favore di questo provvedimento, che consegue l'obiettivo minimo che doveva necessariamente prefiggersi: prefiggersi: apportare modifiche alla legge n. 196 del 2009 in modo tale da armonizzare le scadenze della finanza pubblica italiana al nuovo ciclo della *governance* della finanza pubblica stabilito dall'Unione europea, dal Consiglio ECOFIN del settembre 2010, che siamo ormai soliti chiamare il semestre europeo, che entra in vigore dal 2011. Questo obiettivo minimo risponde a un cambiamento di filosofia dell'Unione europea, che passa dalla fissazione di parametri da rispettare e da controllare *ex post*, e quindi da obiettivi di risultato, rispetto al quale controllare gli sforamenti - peraltro senza un'adeguata disciplina sanzionatoria, e se ne sono visti i problemi - a un ciclo di procedure che tendono verso un coordinamento preventivo, non solo delle decisioni di bilancio e delle decisioni finanziarie, ma anche delle politiche economiche e delle riforme strutturali, iscritte in obiettivi di logica pluriennale e con una più adeguata sorveglianza e un più adeguato apparato sanzionatorio. Lo scopo è chiaramente quello di scongiurare crisi finanziarie come quelle alle quali abbiamo assistito in questi anni e intervenire non più solo sui sintomi, ma coordinando insieme le terapie per tali crisi. Naturalmente ciò significa che nei prossimi anni la valutazione delle politiche economiche degli Stati membri sarà fatta prima dell'approvazione da parte dei Parlamenti, in modo tale che gli obiettivi dell'Unione europea possano essere integrati e ricompresi nelle politiche nazionali. Si tratta di un grande passo avanti, da cui può dipendere la sopravvivenza stessa, o quanto meno l'efficacia dell'integrazione

(DFP) e contiene gli schemi del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, oltre a tanti altri elementi previsionali andando a ritroso, entro marzo deve essere indicata una procedura di concertazione con le altre amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali.

poi una serie di adeguamenti sulle scadenze e sui contenuti, di cui si è ampiamente parlato nel dibattito. Questo è il punto da cui si parte. Esso contiene, come ha illustrato il presidente Azzollini, diversi elementi positivi, le modifiche di cui abbiamo parlato inscrivono gli obiettivi in un'ottica di medio termine e introducono novità rispetto alla legge approvata recentemente, nel 2009, per cui ad esempio il risparmio pubblico eventualmente conseguito potrà essere utilizzato per coprire riduzioni di entrata - e non maggiori spese - e a condizione che il saldo sia positivo (si tratta dunque di un divieto implicito di aumentare la spesa corrente con l'eventuale risparmio pubblico). Le maggiori entrate, rispetto alle previsioni, potranno essere utilizzate solo per migliorare i saldi e non per coprire

adeguatamente considerate nel documento di aprile. Va detto, però, che per molti aspetti il bicchiere può essere anche considerato mezzo vuoto: tra due giorni il vertice dell'Unione europea deciderà su alcuni elementi fondamentali, come il fondo di stabilizzazione anticrisi

improduttiva, passando dalla filosofia dei tagli lineari a quella dei tagli selettivi e della riqualificazione della spesa pubblica. Quindi, occorrono riforme strutturali nei maggiori comparti della spesa pubblica, secondo le indicazioni della stessa Unione europea (che noi troppo spesso

di servizi pubblici che non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli dei primi due, e di alcuni altri Paesi in classifica. Tanto meno sarà possibile traguardare una riduzione delle tasse per le famiglie, che consentirebbe più reddito per i consumi e quindi rappresenterebbe una buona mossa verso la ripresa, e delle tasse per le dunque, è necessario, ma non è sufficiente, ed anche per questo abbiamo votato a favore di molti emendamenti presentati; tuttavia non possiamo e non intendiamo cadere nella tentazione del "benaltrismo". Possiamo affermare che con questo provvedimento poniamo le basi minime dal punto di vista tecnico, sapendo che sarà necessario, di fronte alle nuove sfide politiche dell'Unione europea, impostare una diversa costruzione delle nostre politiche finanziarie. L'Italia è stata una pioniera della

la "madre" di una seria riforma di contabilità, che è la certificazione dei bilanci da parte di un'istituzione pubblica, esterna o interna al Parlamento.

fare riferimenti evangelici): una costruzione senza la pietra d'angolo, per quanto l'architettura possa essere gradevole, piacevole e solida, manca del punto di appoggio di riferimento.

Ebbene, alle società private si impone, nel caso della certificazione, un atto dovuto, per chiarezza trasparenza e rispetto di quell'articolo della Costituzione che prevede che il risparmio sia salvaguardato e garantito. Quando però questo risparmio fa riferimento ai bilanci delle pubbliche amministrazioni, la certificazione non c'è. non c'è. Nonostante l'entità consistente della capitalizzazione delle società private in Borsa, l'entità di cui stiamo parlando e rispetto alla quale non c'è alcuna certificazione (come abbiamo vissuto tutti nelle esperienze quotidiane e settimanali in quest'Aula), quest'Aula), rappresenta un bilancio di 812 miliardi di euro all'anno dal lato della spesa, cento circa del prodotto interno lordo, e dal lato delle entrate stiamo parlando di circa 740 miliardi di euro all'anno, circa il 47 per cento del prodotto interno lordo. Questo è l'andamento costi-ricavi, il conto economico, rispetto al quale, per le società quotate, giustamente, c'è l'obbligo della certificazione, mentre per questa entità, che rappresenta la metà del reddito prodotto da tutti gli italiani, rimaniamo nel vago. Ma c'è una motivazione politica nel volere questo. Non credo che i 127 senatori che hanno votato contro il precedente emendamento lo abbiano fatto solo per una non piena conoscenza o consapevolezza: l'hanno fatto correttamente per rispondere all'indicazione data dal loro Governo. Quindi, da questo punto di vista, è stato un voto di coerenza rispetto alle indicazioni del Governo. Ma quello che voglio sollevare in quest'Aula è questo punto: punto: un Governo che apparentemente vuole perseguire il rigore finanziario, sembra paradossale ed assurdo che esprima parere contrario nel porre la pietra d'angolo nella riforma della legge di contabilità e nel suo attuale adeguamento alle normative europee. Ebbene, signor Presidente, cari colleghi, non è un paradosso. È la chiave vera per capire la strategia della politica economica italiana di questi anni, cioè la deviazione dell'attenzione di tutti esclusivamente verso i saldi di finanza pubblica, cui l'attenzione è posta esclusivamente alla differenza tra le entrate e le spese, il *deficit* e il debito. Ovviamente questa attenzione è sacrosanta per salvaguardare gli equilibri finanziari; ma non è la politica economica, perché uno stesso *deficit* e di conseguenza uno stesso debito può provenire da 100 di entrate e 110 di spesa oppure da 1.000 di entrate e 1.010 di spesa. Il saldo, la differenza, sarebbe sempre 10, ma tutti possono capire che la realtà economica e della politica economica è radicalmente diversa se entrate e spese si aggirano intorno a 100 oppure attorno a 1.000, a parità di saldo. Perché Perché questo? Perché l'apparente perseguimento del rigore sui saldi consente di nascondere i giochi delle tre carte sulle componenti di entrata e di spesa, consente ad una burocrazia autoreferenziale e ad una politica connivente di giocare sui numeri facendo apparire il saldo in un certo modo ma senza dire che il risultato in termini di saldo può avere al suo interno duemila soluzioni diverse. Lo verifichiamo ogni volta: quando c'è la volontà politica di trovare 10, 20, 50 milioni di euro, questi appaiono come funghi la mattina dopo l'alba, mentre quando non c'è volontà politica si risponde che non c'è più un euro. Siamo nella totale discrezionalità della politica economica, rispetto alla quale le Aule parlamentari, e direi quasi tutti i componenti del Consiglio dei ministri, non hanno la piena consapevolezza delle scelte economiche e di politica economica che vengono compiute. E allora, questo non è rigore finanziario: è uno specchietto per le allodole.

Nel corso degli anni tante volte, oltre al sottoscritto, molti altri colleghi sono andati a vedere i documenti ufficiali della finanza pubblica: lo accennava un minuto fa il collega Musso. Ebbene, se prendete i documenti di finanza pubblica degli ultimi dieci anni, vi accorgerete che cambiano di anno in

- ciò significa che c'è una volontà politica di mantenere il monopolio dei numeri nella inconsapevolezza frequente delle Aule parlamentari e di molti componenti dello stesso Governo rispetto alla politiche che si decidono. Un'ultima osservazione, signor Presidente, cari colleghi: in queste condizioni, fra poche settimane dovremo affrontare il nuovo Patto di stabilità europeo. Ci si rende conto che, almeno teoricamente, per come è scritto il Patto, all'Italia si chiede, sui saldi, una manovra di 45 miliardi di euro l'anno per i prossimi anni?

se c'è uno al comando che sa tutto, affidiamo tutto a quell'unico che ha il comando. Il mio dubbio è che spesso quell'uno al comando non sappia tutto, e qualche volta sappia ben poco.

Oppure possiamo parlare di crescita inclusiva, ossia del campo riguardante gli aspetti della coesione sociale e territoriale. Queste tre grandi priorità, che compongono anche

si sono confrontate, e magari scontrate, posizioni assolutamente differenti sullo stesso argomento da parte di esponenti diversi,

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, economica dell'Unione europea, questo provvedimento ha assunto un significato politico e un rilievo normativo ben più consistente rispetto alla situazione di partenza dell'*iter* legislativo. La recentissima intesa, basata su un pacchetto di sei misure legislative europee, tra cui la riforma del Patto di stabilità anti-*deficit* e le nuove procedure di debito eccessivo, sarà con ogni probabilità - come ci è noto - approvata dai Capi di Stato e di Governo dell'UE nei prossimi giorni e dal Parlamento europeo

e l'aggiustamento dei conti verso il pareggio del bilancio, l'obiettivo di riduzione graduale ma costante del debito pubblico eccedente il 60 per cento del PIL nella misura - come sappiamo - di un ventesimo all'anno a partire dal 2015, dato che sarà considerato come *benchmark* numerico per il ritmo di discesa dei debiti che superano la soglia suddetta, nonché l'introduzione di meccanismi sanzionatori semiautomatici, l'incremento del fondo anticrisi fino a 500 miliardi di euro, una procedura preventiva di allerta Non so se il giudizio più adeguato per l'intesa raggiunta sia quello espresso dal nostro Ministro dell'economia, secondo il quale si tratterebbe di una buona intesa per l'Italia, l'unica possibile, o quella critica del capo della BCE Jean Claude Trichet, secondo il quale il rafforzamento della *governance* è insufficiente per far fronte in futuro in modo efficace ad eventuali crisi dell'euro. Ciò che è certo è che il nostro Paese, al pari degli altri e più degli altri, dovrà sempre più adeguare la propria politica economica e di bilancio agli obiettivi stringenti fissati in sede europea e ciò dovrà fare sia sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle manovre finanziarie e degli interventi di riforma strutturali, che osservando le procedure di valutazione *ex ante* dei provvedimenti adottandi in corso d'anno, di osservazione durante il semestre e di controllo *ex post* degli interventi adottati. Dunque, un'ulteriore quota di sovranità economica e finanziaria, dopo l'introduzione dell'euro, viene ceduta all'Europa in cambio di un costante dialogo istituzionale che non riguarderà soltanto i Governi ma anche il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali. È dentro tale contesto che va collocato l'intervento di modifica della legge di contabilità, che pure avevamo riformato insieme circa un anno e mezzo fa. L'*iter* di riforma della legge di contabilità è iniziato qualche mese fa, come è noto, alla Camera con un'iniziativa legislativa parlamentare congiunta della maggioranza e dell'opposizione. Il lavoro alla Camera, certamente proficuo, concluso con un voto unanime, si è sviluppato soprattutto sulla modificazione della tempistica e di taluni contenuti degli strumenti della sessione di bilancio, che inizia a primavera e si conclude a fine anno dentro le nuove regole di controllo e di dialogo preventivo e successivo con l'Unione europea. L'esame del provvedimento, però, non ha tenuto conto alla Camera (e non poteva tenerne conto per ragioni temporali) dell'esatto contenuto dell'intesa definitiva raggiunta in sede europea. In questo ramo del Parlamento, quindi, i termini del confronto sono mutati. I punti di dissenso con il Governo e la maggioranza muovono da due novità emerse dopo la prima lettura alla Camera. Innanzitutto, il contenuto dell'accordo dei Ministri dell'ECOFIN dell'11 marzo scorso impegna gli Stati a scegliere uno specifico strumento normativo nazionale purché la normativa recettiva della nuova *governance* europea «abbia una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte». Ciò con riferimento alla necessità di garantire la disciplina di bilancio nazionale a mezzo di regole che realizzino appunto, in modo vincolante, un «freno all'indebitamento», regole collegate al saldo primario o regole di spesa. Insomma, l'Unione europea ci dice: fate come ritenete più opportuno, ma gli obiettivi devono essere garantiti attraverso norme cogenti, a prescindere dal loro rango». Sappiamo che altri Paesi stanno operando in modo efficace in tale direzione, ad esempio la Francia, con modifiche costituzionali, come ci ha ricordato il collega Morando in data di ieri. Con l'aiuto del collega Ceccanti disponiamo, signor Presidente, del testo del *projet de loi constitutionnelle* presentato da una certo signor Sarkozy all'Assemblea nazionale di Francia in data 16 marzo 2011, cioè cinque giorni dopo la sottoscrizione dell'accordo in sede europea: così operano luogo, l'emendamento approvato in Commissione bilancio, confermato in Aula, depotenzia sostanzialmente il passaggio al bilancio di cassa già previsto nella riforma del 2009, la cui piena attuazione avrebbe consentito un più efficace ed effettivo controllo dei flussi di spesa e il graduale superamento dell'abnorme accumulo di residui passivi ed attivi. L'abbandono sostanziale, per effetto della innovazione apportata in Commissione, di tale importante novità contabilistica attenua fortemente gli obiettivi della trasparenza e della responsabilità nella gestione dei nostri conti pubblici. A tali novità si aggiunge la persistente contrarietà, registrata anche questa mattina, le cui motivazioni continuano ad essere insediate fuori dalle Aule parlamentari, al rafforzamento degli strumenti e delle strutture tecniche di gestione delle basi informative e valutative dei nostri conti pubblici a mezzo dell'integrazione dei Servizi del bilancio di Camera e Senato o con altro strumento o autorità. Queste sono le ragioni del nostro dissenso, signor Presidente, per larga parte sopravvenute alla prima lettura della Camera e l'esame dell'Assemblea non ha consentito di superarlo, nonostante le nostre proposte precise e ragionevoli, molto ben illustrate e sostenute dal relatore di minoranza, senatore Morando, e dagli altri colleghi intervenuti, che voglio ringraziare per il lavoro svolto. Signor Presidente e onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un passaggio storico, non soltanto per l'integrazione dell'area dell'euro, ma per il grado di responsabilità che la politica italiana dovrà esercitare nei prossimi anni essendo obbligata a percorrere, a ritroso ed in salita, la difficile via del risanamento dei conti pubblici. Il debito pubblico italiano è il primo in Europa e il terzo in termini assoluti al mondo. Il suo ammontare, che a gennaio del 2011 ha raggiunto il nuovo *record* di 1.879 miliardi di euro, è per oltre la metà nelle mani di investitori stranieri. Nei prossimi 24 anni dovremo tornare al livello del 1975, trentasei anni fa. Sì, il rapporto tra il debito e il prodotto era al 60 per cento nel lontano 1975 e lì dovremo tornare. Da allora il debito è cresciuto mediamente di un 5 per cento all'anno, ed anche più, fino al 1994, quando toccammo il livello massimo per cento del PIL, per poi iniziare una discesa lenta ma graduale negli anni successivi, con una significativa coincidenza: salvo rare eccezioni, durante gli anni di governo del centrosinistra il rapporto debito-PIL è sceso, durante gli anni di governo del centrodestra il debito è tornato a crescere, come è accaduto, certo anche per effetto della crisi, negli ultimi anni, con una crescita del debito in tre anni di circa 15 punti. È impressionante, al riguardo, signor Presidente, analizzare la tabella di evoluzione del debito pubblico in Italia dagli anni '70 ai giorni nostri: dati che ci dicono molto di più di ogni altro argomento propagandistico su quanto è accaduto nella storia del nostro Paese negli ultimi 40 anni. Le regole devono, secondo noi, riflettere tale percorso risanatore che gli errori del passato ci costringono a seguire. Tale eccezionale impegno dovrà coesistere con quello, anch'esso contemplato nella nuova costituzione economica europea, che ci chiede di adottare misure di stimolo per la competitività e l'occupazione, in particolare giovanile e femminile, oltre che volte a rafforzare la stabilità finanziaria. Tommaso Padoa-Schioppa, Signor Presidente, economista e uomo politico italiano ed europeo di rarissima lucidità ed efficacia, che voglio qui ricordare e citare, disse in quest'Aula il 3 ottobre del 2007: «Per troppi anni è stato commesso l'errore di affrontare i problemi dell'oggi ipotecando le risorse del domani, per troppo tempo è sembrato che la saggezza e la bravura consistessero, come in un rodeo di cavalli, nel restare in sella rinunciando a darsi una direzione». Restare in sella rinunciando a darsi una direzione: sembra una metafora sul tempo presente, applicabile anche a questa discussione. La direzione giusta e peraltro corrispondente a precisi impegni assunti in sede europea dal Governo nella sua massima espressione deve essere, secondo noi, quella dell'individuazione di strumenti, strutture, supporti normativi certi e cogenti per garantire il più eccezionale degli sforzi e delle responsabilità richiesti alle classi dirigenti dell'oggi e del domani. Voi, signori del Governo e della maggioranza, avete scelto un profilo basso, sostanzialmente o potenzialmente elusivo degli obblighi di recente assunti in sede comunitaria. Avremmo voluto fortemente votare a favore di questo provvedimento per consentire al nostro Paese di presentarsi nel migliore dei modi al nuovo appuntamento con l'Europa. Non possiamo farlo per tutte le ragioni che abbiamo sostenuto sostenuto durante la discussione. A malincuore, quindi, ma forti dei nostri convincimenti, che cercheremo di far valere anche in futuro, dichiaro il voto contrario del mio Gruppo.

colleghe e colleghi, con l'approvazione delle norme sulla contabilità dello Stato ricomprese nella legge n. 196 del 2009, l'ordinamento aveva conosciuto una profonda innovazione rispetto allo schema consolidato applicato per numerosi anni

da legge finanziaria a legge di stabilità - ma anche di carattere sostanziale, in vista dell'adeguamento della funzione parlamentare di indirizzo e controllo sulla gestione della contabilità pubblica alle esigenze di flessibilità e di elasticità richieste dai tempi attuali. A distanza di poco più di un anno da quel passaggio siamo nuovamente chiamati a intervenire nel merito. Non si modifica, in ogni caso, l'impostazione originaria. In sostanza, l'introduzione a livello di Unione europea di una nuova procedura che tende ad un coordinamento più stringente *a priori* delle politiche economiche e finanziarie dei singoli Paesi-*partner* impone la necessità, e anche l'urgenza, di intervenire sui tempi e sulle modalità di programmazione della vigente normativa, allo scopo di armonizzarla pienamente con le regole comunitarie. I cambiamenti della tempistica da seguire nella predisposizione e nell'esame dei documenti di finanza pubblica sono, dunque, finalizzati ad adeguare le procedure nazionali agli obblighi previsti nel semestre europeo. In particolare, la trasmissione del Programma di stabilità alle autorità europee entro il 30 aprile

viene richiesta l'elaborazione per il periodo di programmazione delle previsioni macroeconomiche di finanza pubblica, con la valutazione dei dati tendenziali per il conto economico e con i conti di cassa delle amministrazioni pubbliche, articolate per sottosettore istituzionale. Bisogna essere coscienti che, considerato il calendario in cui gli enti preposti come - ad esempio - l'ISTAT possono diffondere i dati sulla produzione e sul tasso di crescita del PIL, è inevitabile che ciò comporti talune criticità. Occorrerà che tutti i comparti della pubblica amministrazione, compreso il sistema delle Regioni e degli enti locali, acquisiscano una tempistica nella redazione dei documenti contabili e di bilancio in grado di permettere l'acquisizione di dati tempestivi su cui si possano fare previsioni attendibili. Il Programma di stabilità da presentare in sede europea diviene dunque l'asse portante della programmazione economica e finanziaria che il Parlamento esamina e valuta prima dell'invio alle istituzioni economiche. Il Programma, dunque, viene sostanzialmente a sostituirsi alla decisione di finanza pubblica. Completamente nuovo, almeno nella configurazione ora proposta, è invece un secondo documento, un secondo strumento di programmazione europea, il Programma nazionale di riforma, che certo già in precedenza era stato presentato dal Governo alle Camere, in attuazione sia della strategia di Lisbona sia della strategia Europa 2020 e al quale il codice di condotta europea attribuisce invece adesso una assai maggiore concretezza, innestando le riforme finalizzate allo sviluppo e alla crescita dell'economia nella programmazione finanziaria. Entrambi tali documenti, il Programma di stabilità e il Programma di riforma, confluiranno nel Documento di economia e finanza, che sarà completato da una terza sezione volta a fornire alle Camere una più approfondita analisi degli andamenti tendenziali e di finanza pubblica, con riferimento al successivo triennio, al conto economico e al conto di cassa delle amministrazioni pubbliche. Anche in relazione alla tempistica ristretta cui si accennava in precedenza, appare quanto mai opportuno e auspicabile che il Parlamento, in particolare attraverso l'attività delle Commissioni, possa avere sin dalla fine del mese di gennaio occasione di discussione e di analisi, confrontandosi con le istituzioni europee, al fine di chiarire gli indirizzi politici di fondo e i contenuti degli atti di programmazione. Spetterà quindi alle Camere, e in particolare alle Commissioni, adottare un nuovo metodo di lavoro più sistematico, incentrato sull'attività di controllo e di indirizzo e strettamente coordinato con i processi decisionali dell'Unione europea, in modo da poter seguire ed orientare l'attività di programmazione economica e finanziaria. Si creano dunque le condizioni per una più evidente sinergia tra gli organi legislativi nazionali ed europei che consentirà alle Camere, congiuntamente al Parlamento europeo, di svolgere un ruolo più pregnante nell'identificazione delle strategie unitarie e della programmazione economica e finanziaria, allo scopo di rafforzare la capacità di risposta dell'intero sistema Europa alle sfide della globalizzazione dei mercati. Le modifiche introdotte dalla legge n. 196 del 2009 si presentano come necessario adeguamento e miglioramento delle regole previste per la contabilità pubblica, confermando quindi l'impianto originario, teso a liberare i documenti di bilancio dall'appesantimento cui erano andati incontro negli anni precedenti, fino a comportare mesi e mesi di lavoro delle Camere. Ricordo che il punto di svolta rispetto a questo stato di cose è arrivato con il Governo Berlusconi, dal 2008, e con la legge finanziaria 2009 - o l'anticipazione della legge finanziaria 2009 - con la fissazione mediante il decreto-legge n. 112 del 2008, dei saldi di bilancio entro cui muovere le previsioni, ponendo severi limiti alla manovra di bilancio. In tale prospettiva, la legge n. 196, con le attuali modifiche, si figura come una sistematizzazione ed una formalizzazione stabile delle decisioni assunte all'avvio della legislatura dal Governo e, quindi, delle decisioni di interpretare il tema della finanziaria e del bilancio in modo assolutamente discontinuo rispetto alla prassi invalsa negli ultimi anni. Si rafforzano dunque i presupposti affinché il Parlamento possa concentrarsi sulle funzioni di programmazione e di indirizzo in modo pieno, senza invadere il campo gestionale tipico dell'Esecutivo, e affinché nel contempo allo stesso Parlamento siano forniti gli strumenti effettivi per un controllo puntuale ed efficace delle politiche e delle scelte realizzate dalle amministrazioni, così come si conviene all'organo titolare della sovranità popolare, migliorando con le modifiche in esame la capacità di raccordo con le decisioni europee. Questo è lo strumento. Molti degli interventi, signor Presidente, colleghi, sono entrati nel merito,

Noi abbiamo rafforzato il doppio bilancio, ma dobbiamo anche ricordarci che, dalla legge n. il sistema politico italiano, il Governo, il Parlamento e tutte le pubbliche amministrazioni hanno ragionato per competenza, ignorando la cassa. Dobbiamo altresì ricordarci che a partire dal 1996 alcune scelte politiche hanno

un vero bilancio di competenza, che quindi abbia la copertura dei costi di competenza con le entrate di competenza, e un vero bilancio di cassa che tenga conto dei flussi finanziari. Quindi, non copriamoci con lo strumento: lo strumento è una funzione per entrare nel merito. Questo, per permettere al nostro Paese anzitutto di svolgere un ruolo attivo in ambito europeo ed essere parte attiva

impoverire i privati per far diminuire il debito pubblico: la crisi ci ha dimostrato che sono un tutt'uno e che non cambiano i saldi. Servono invece azioni di riforma,

sia nell'interesse di tutte le forze presenti in Parlamento la condivisione di regole valide e chiare in un settore di così grande rilevanza come la contabilità e la finanza pubblica ed esprimo quindi il pieno sostegno e il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.

Un attimo, perché sono d'accordo con il vice presidente Chiti nel chiedere ai colleghi,

supera le criticità di natura economica che avevano suscitato alcune perplessità in sede di approvazione da parte del Consiglio dei ministri. da parte del Consiglio dei ministri. Con il testo che verrà fuori dall'approvazione degli emendamenti della Commissione sono state previste tutte le ipotesi che possono interessare

potrebbero essere tenuti a pagare una giornata di lavoro senza un'opportuna e corrispondente controprestazione.

Non possiamo che compiacerci che il Governo, nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, abbia individuato questa data come un giorno festivo, direi a tutto campo, perché già in un precedente provvedimento era stata prevista la festa del 17 marzo 2011, ma non erano stati disciplinati gli effetti sostanziali e, in particolare, quelli economici, che derivavano

a tutti gli effetti. Credo che sia stato importante, anche per chi al momento può aver avuto qualche dubbio sulla scelta governativa, che questa discussione venga fatta in Aula successivamente alla celebrazione del 17 marzo scorso, perché in quell'occasione si è fatta giustizia di tanti pregiudizi e, soprattutto, si è dato campo ad una presenza istituzionale e, in particolare, quella del Capo dello Stato, al quale siamo grati, che ha saputo dare un taglio davvero unitario alla celebrazione di questa data fondamentale per l'Italia e per il suo futuro, oltre che per il suo passato, coniugando i valori del passato con le prospettive del presente e del futuro. Il Capo dello Stato, soprattutto nella cerimonia di Montecitorio, con una vera e propria *lectio magistralis*, ha saputo darci una lezione di come si approfondiscano e si valutino, anche con spirito critico, le vicende del passato, senza rinunciare ai valori che da esse emergono. Ritengo che questo sia il dato più significativo, che dovremmo apprendere

che oggi sta decollando e che non contraddice l'Unità d'Italia: semmai contraddice il centralismo che fino ad ora ha purtroppo caratterizzato il nostro Paese. Il centralismo non è solo quello di Roma, ma può essere anche quello delle varie capitali regionali, e di esso dobbiamo sempre diffidare. Essere contrari al centralismo significa essere favorevoli alla

Ritengo che questa giornata particolare e la decisione di farne una grande festa nazionale, una festa di popolo

sia stata molto opportuna. Le ragioni che l'hanno motivata hanno trovato già una risposta convinta nella partecipazione di popolo, così vasta, positiva e convinta da parte dei cittadini italiani, in tutte le parti del nostro Paese, che è andata al di là

di davvero popolare, contro ogni rischio di retorica patriottarda, da un lato, e di banalizzazione celebrativa, dall'altro.

alcune. Le parole del Presidente della Repubblica, che ha richiamato anche il relatore, hanno detto chiaramente che il Paese sta attraversando un periodo di difficoltà sul piano economico e sul piano della necessità di trasformazioni istituzionali - non certo ultima quella del federalismo nei suoi diversi aspetti - e che uno dei problemi che attanagliano la società italiana, collegato alle difficoltà economiche, da un lato, e alle riforme istituzionali, dall'altro, è quello

perché, insieme ad altri di battaglia e di indipendenza, cioè di guerra contro un nemico, un oppressore, un invasore - e quindi, la bandiera dell'indipendenza nazionale e della libertà del popolo italiano hanno sempre contenuto anche elementi di emancipazione sociale, di avanzamento e di progresso. I grandi democratici che hanno fatto il Risorgimento chiedevano libertà, unità e Costituzione. I valori messi in campo dai repubblicani in modo più avanzato, ma anche dal pensiero liberale più moderato, nella richiesta di Costituzione, erano

A Milano tutti gli anni festeggiamo insieme le Cinque giornate di Milano. Non sto neanche a citare i nomi di Cattaneo, Confalonieri, Cavour, Mazzini, Garibaldi, lo stesso Gioberti e le donne. Scusatemi una parentesi per ricordare che, come sempre, nelle fasi rivoluzionarie di trasformazione le donne sono protagoniste; poi, quando magari un po' di restaurazione, gli uomini tendono a rimetterle al loro posto,

che hanno fatto il Risorgimento, qualcuna anche armata e qualcuna con un'opera di accompagnamento che è stata fondamentale.

l'«Inno al re» e usare come mito storico la romanità, la Lega preferisce dei feticci fasulli come i riti celtici e le polle d'acqua, quando avrebbe lì, a casa sua,

di riuscire ad essere contemporaneamente una buona milanese, una buona italiana e, se permettete, anche una coerente federalista. Signora Presidente, onorevoli colleghi, lo ha accennato anche la collega Adamo in apertura, con delicatezza: ci sono due riserve che che non possiamo fare a meno di considerare nello svolgere questo ragionamento sul provvedimento in primo luogo, il provvedimento è stato proposto come decreto-legge con ragioni di necessità e di urgenza al riguardo di un anniversario datato 150 anni fa. Si poteva davvero invocare i criteri di necessità ed urgenza per un caso di questa natura? In realtà il decreto in quanto tale nasce da inadempienze imputabili alla prassi del Governo legislatore.

I dubbi interpretativi che nascevano da questa norma hanno indotto l'Esecutivo ad adottare, 22 giorni prima della festa, un decreto per dichiararne gli effetti civili. è abbastanza paradossale che si possano invocare ragioni di necessità e urgenza per assicurare la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo, e solo per il 2011, giorno festivo a tutti gli effetti civili. La seconda riserva riguarda il fatto che ormai stiamo discutendo di tale questione con un ritardo di qualche giorno.

convertire questo decreto‑legge in tempo, entro il 17 marzo, e garantire in questo modo un corso direi naturale delle cose? Invece stiamo convertendo

Viene il dubbio che in questa procedura così strana abbia in un certo senso imposto una ragion d'essere una certa voglia di trascuratezza, di disinteresse per la ricorrenza, che all'interno del contesto della maggioranza si è avvertita in maniera palpabile. L'emendamento introdotto in Commissione non ha nulla di forzato: mira semplicemente a sottrarre

riguardo a costruzioni di nuove feste nazionali, intende evidenziare che, se questa ricorrenza deve essere celebrata, non si capisce perché si debba limitare la volontà

ai lavoratori e a tutte le persone attive della società italiana il ricordo del momento in cui il crogiuolo dell'Unità d'Italia ha trovato una sua solidificazione. Sulla connessione tra spirito risorgimentale e spirito della Resistenza conto di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

credo di dire quello che molti colleghi, forse tutti, possono dire se hanno frequentato le nostre sedi, i nostri paesi, là dove abitiamo, dove siamo eletti, e hanno visto l'entusiasmo che c'è stato attorno a quella che è stata considerata una festa quasi personale. Avendo parlato a lungo con studenti in diverse scuole, e qualche volta di sera con gli studenti e le loro famiglie,

non solo ricordando le patriote lombarde - mi vengono in mente le venete, come la Serego Alighieri e la Avesani - c'è un fatto che caratterizza la storia di tutta la vicenda umanitaria nel mondo. In Italia, tra Solferino e San Martino, durante la Seconda guerra di Indipendenza è avvenuto un fatto che ha segnato la storia del mondo.

le donne di Castiglione delle Stiviere e di altri paesi vicini, utilizzando secchi d'acqua e lenzuola strappate, hanno creato bende, hanno guarito, sanato, aiutato e coperto i morti, senza guardare alle giubbe e alle bandiere. I feriti in guerra erano solo uomini.

Presidente, onorevoli colleghi, pensate che gli uomini sono riusciti a mettere limiti anche alle guerre. Il diritto internazionale umanitario si chiama anche diritto dei conflitti; è fondato sulle Convenzioni di Ginevra, sui Protocolli aggiuntivi di Vienna e su quelli che stanno ancora adesso nascendo in ragione del fatto che stanno profilandosi nuovi crimini contro l'umanità. crimini di guerra, come lo stupro perpetrato contro le donne in termini di genocidio. Siamo il Paese che può gloriarsi di essere la culla del movimento di volontariato umanitario più grande al mondo, la Croce rossa.

che copre tutta l'umanità nelle difficoltà, non ci fa velo essere orgogliosi anche della nostra bandiera. Abbiamo visto quanto il tricolore sia stato sventolato, non solo dopo le affermazioni sportive, perché ciascuno se ne è sentito coperto. allora associarmi a chi ha pensato che questo 17 marzo potrebbe essere una festa per sempre. Penso al 4 luglio per gli americani: un grande Paese federalista trova nella festa dell'unità il momento in cui celebra anche la storia con cui si è aggregato fino a diventare una grande federazione. È il 4 luglio che conta, le 50 stelle nell'azzurro e le strisce, che ricordano che lì sotto ci sono tutti gli americani. Di conseguenza, insultare la bandiera o chiedere che sia usata per usi non consentiti è un delitto, perché è un delitto contro ciascun americano. Il 17 marzo ho capito che anche noi siamo riusciti a inculcare questi pensieri. Abbiamo una storia, che si è dipanata in 150 anni e che ci sta dando messaggi e lezioni per il momento presente. Questo nostro Paese ha in mano il simbolo della Croce Rossa insieme alla bandiera. Apparteniamo alla NATO

Nel 1977 la legge intervenne a ridurre, da 16 a 10, le festività obbligatorie, sulla base di un accordo interconfederale; e lo fece senza introdurre compensi sostitutivi. Il compenso sostitutivo venne introdotto da quello stesso accordo interconfederale cui la legge dava attuazione, ma Il permesso sostitutivo, retribuzione aggiuntiva sostitutiva della festività soppressa, conserva dunque come unico fondamento giuridico l'accordo collettivo. Altrettanto, poi, è avvenuto per il settore del pubblico impiego; e qui è evidente che il provvedimento in discussione nasce da una preoccupazione riferita soprattutto all'esigenza di

a un obbligo di retribuzione aggiuntiva per la festività soppressa del 4 novembre che, in realtà, non è previsto dalla legge; e poiché l'accordo interconfederale,

ci può essere qualche azienda che per difetto di iscrizione a Confindustria o ad altra associazione imprenditoriale firmataria resti fuori dall'area di applicazione della norma collettiva. sembra che, secondo logica, si debba intendere la norma che stiamo adottando, nel caso in cui l'accordo interconfederale non si applichi, come fonte originaria di un obbligo retributivo per il 17 marzo. Tuttavia, la formulazione letterale della norma per questo aspetto è difettosa perché

due considerazioni: la prima di carattere tecnico, la seconda di carattere politico e storico. Come è noto, i Ministri della Lega Nord avevano sollevato delle perplessità in relazione alla copertura di questo provvedimento,

dalla motorizzazione di massa (dunque, ancora la FIAT, ma non solo), dalla televisione che divulgava un senso di benessere e, di sviluppo e dell'inizio del *boom* economico e della fortuna del nostro Paese. E adesso siamo a 150 anni

Pensiamo che un'idea forte possa e debba essere proprio questo benedetto federalismo, non solo perché l'Europa ci impone il rigore dei conti pubblici, ma perché abbiamo davvero bisogno di dare una scossa all'Italia, non solo per l'economia ma soprattutto per trovare un motivo serio per stare insieme e per dare sviluppo al nostro Paese. Prima si citavano grandi Nazioni: gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, la Svizzera; tutti Stati, soprattutto questi ultimi, federali, che, quindi, stanno molto bene insieme, nelle proprie diversità. Noi pensiamo che questa possa essere davvero l'idea forte per questo Paese. Dopo 150 anni, al di là di pura retorica, che poi lascia il tempo che trova, l'idea forte può essere proprio questa del federalismo fiscale e, non solo: anche del federalismo politico, che è la sfida successiva. Grazie, Presidente,

Ci sono state manifestazioni di ogni tipo, di ogni carattere, per le strade, per le piazze. Credo però ci sia stato un clima generale di condivisione, un clima gioioso. Abbiamo visto anche con quanta emozione i nostri concittadini si sono stretti intorno ai nostri simboli, l'Inno d'Italia, le bandiere, al di là dell'enfasi, con un riconoscimento di amore per la propria terra e per la propria storia

Sì, è stato un momento per riconoscersi, per ritrovarsi, forse anche più forte ora, perché siamo tutti molto smarriti per tante e tante vicende, nazionali, internazionali, anche epocali,

molto lontani; ci si sente tutti più soli. Ritrovare, quindi, un'identità, che non è nazionalismo ma che è un nuovo patriottismo consapevole, forse anche con qualche punta di amaro, ma un patriottismo voluto, considerato necessario, importante. Qui tornano due grandi parole che il Presidente della Repubblica ha pronunciato, anche cogliendo ed interpretando, credo, lo spirito del popolo italiano: orgoglio e fiducia, al di là dei luoghi comuni, al di là della retorica. Sì, c'è bisogno oggi di orgoglio e di fiducia, ma anche di coraggio con il quale dovrebbe agire una classe dirigente che rinsalda i propri legami con la comunità, che sa indicare un cammino, una prospettiva, proprio in queste prove così difficili, non dimenticando le grandi difficoltà che vive il nostro Paese. A 150 anni dall'Unità d'Italia, dopo il Risorgimento, le guerre, il fascismo, la Resistenza, la Guerra fredda, il terrorismo, l'Europa e la globalizzazione, ricordiamo le tappe più importanti: i primi 50 anni, quando con orgoglio l'Italia si avviava verso un progresso economico e da un Paese agricolo diventava un Paese industriale; il 1961, i 100 anni, quando il *boom* economico faceva dell'Italia un Paese al secondo posto nel mondo in termini di crescita del PIL, dopo il Giappone, quando il Governo si apriva alle forze di centrosinistra per affrontare riforme strutturali come la nazionalizzazione dell'energia elettrica o la riforma della scuola media,

meridionale. È indubbio il contributo che il Sud ha dato alla forte crescita del sistema Paese, a cominciare dalle risorse che le banche del Nord hanno drenato dal 1880 al 1925 dai 5 milioni di migranti meridionali che dal 1950 al 1980 hanno costruito questo Paese. Già nel 1900 Saverio Nitti ricordava e mobilitava le coscienze e l'opinione pubblica nazionale e Sud, dimostrando il costante trasferimento di risorse dal Sud al Nord del Paese. I suoi ragionamenti

venduti nel mercato del Sud; senza combattere la mafia e la camorra nel Mezzogiorno non si potrà combatterle anche nel resto del Paese. Ecco, una nuova sfida: ricercare insieme in un momento di crisi come andare oltre, Forse il federalismo può essere un riequilibratore, ma non può essere un separatore. O cresciamo tutti o non cresciamo. Questa maggioranza che aveva grandi potenzialità

per superare egoismi e particolarismi nell'interesse del Paese. L'Italia ha bisogno di guardare al futuro per i suoi giovani, per le nuove generazioni che non avranno la vita dei propri padri e che soffrono tantissimo per il problema del lavoro, dell'occupazione,

perché ognuno ha fotografato una parte di una verità complessa e articolata della quale, però, dobbiamo saper cogliere i valori fondamentali e ciò che oggi rimane nelle nostre coscienze.

che si era ritenuto, probabilmente senza un approfondimento, che fosse sufficiente questa indicazione per avere, in qualche modo, chiuso la questione della festività nazionale. In realtà, ci si è poi resi conto che le ricadute economiche sul settore pubblico e sul settore privato erano tali da richiedere alcune precisazioni, che sono state inserite in questo decreto-legge e, ancora di

definitivamente), di ricomprendere tutte le vicende complesse e articolate che riguardano le ricadute di tale festività fissata per il 17 marzo, ancorché per il solo 2011. Per quanto riguarda

una regolamentazione di carattere economico, alla quale fa riferimento il testo del decreto-legge, che non priva i lavoratori e i datori di lavoro di nessuna delle loro positività economiche che, invece avrebbero potuto essere messe in crisi dalla previsione di una festività senza un'ulteriore normazione.

Stabilire che la Giornata dell'unità e dell'indipendenza nazionale sia celebrativa e non una festa significa in qualche modo classificare come di serie B detta ricorrenza, la quale invece - a mio sommesso avviso, ma anche grazie all'accoglienza ricevuta sul territorio - meriterebbe comunque una celebrazione di altro livello. Le giornate nazionali sono oramai diventate tantissime. Si assiste ad una proliferazione

a favorire una iniziativa da concludersi entro il 2011, eventualmente anche di carattere legislativo, volta al riordino delle festività nazionali Per quanto riguarda la seconda parte dell'impegno, che entra invece in aspetti più tecnici, e che al limite potrebbe configurarsi come limite della delega al Governo, proporrei di ricostruire questa parte come premessa del suo ordine del giorno. In tal modo il Governo si può impegnare nel suo ruolo, nelle modalità che ho citato prima e lei ha compiutamente espresso, quali sono le indicazioni, le quali però, in relazione alla natura delle iniziative e al ruolo del Governo in questa iniziativa, se legislativa ovvero di carattere regolamentare, potranno trovare più compiuta applicazione. Se riformulato in questo modo, il Governo accetta anche l'ordine del giorno

al rispetto della Costituzione, su cui ricordo che i membri del Governo hanno giurato, mi sembra veramente eccessivamente provocatorio e istituzionalmente poco corretto.

riformulato, di decidere la conferma del Comitato nazionale per le iniziative oppure una sua riorganizzazione, alla luce dell'esperienza, che è certamente riuscita. Voglio ricordare che il testo in questione prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni-Autonomie, la funzione del servizio pubblico radiotelevisivo, la collaborazione della Presidenza del Consiglio e del Ministero per i beni e le attività culturali con i Ministeri dell'istruzione e della gioventù. L'esperienza della celebrazione e delle iniziative collegate è stata certamente molto positiva. Penso allora sia saggio che, monitorandolo in sede parlamentare e in collaborazione con le iniziative parlamentari, il Governo possa valutare se tenere in vita, senza accrescimento di spese, l'attuale Comitato o riformularne il compito d'ora in avanti. In merito all'ordine del giorno G102,

non più come festa che comporta astensione dal lavoro il 4 novembre: ci sono il 25 aprile e il 2 giugno, le due festività relative alla Liberazione e all'istituzione della Repubblica, e ora questa celebrazione straordinariamente riuscita, che, mi permetto di sottolineare, rivolgendomi ai colleghi dell'Italia dei Valori, più che all'indipendenza dell'Italia, che è un concetto francamente discutibile, si richiama alla nascita della Nazione e all'Unità nazionale attraverso ciò che avvenne il 17 marzo 1861.

alla programmazione delle ferie, con riferimento alla prima industria nazionale, che è il turismo, e che dovrebbe essere affrontata, al di là del dibattito che di volta in volta si apre su una celebrazione nazionale, nazionale, con uno sguardo di insieme. Penso ad un'attualizzazione delle festività civili e religiose dentro il calendario nazionale, ad una programmazione delle ferie, ad una programmazione delle ferie, delle vacanze scolastiche (che è competenza delle Regioni), ad un'organizzazione dell'industria turistica, tra le festività estive,

a seconda della stagione turistica. Se voi andate sulla costiera friulana e veneta nei primi dieci giorni di settembre, trovate moltissimi bavaresi, perché la Baviera prolunga le sue vacanze, alternandole in modo da favorire anche la rotazione nelle stagioni sciistiche invernali. È chiaro che è una problematica nazionale, ma anche, in un certo senso, federalista, da organizzare sulla base dei programmi e delle esigenze dei territori, vedendola però in chiave d'insieme.

celebrativa attraverso le scuole, il sistema pubblico radiotelevisivo ed il sistema degli enti locali. È questo un grande compito che la Repubblica,

questo ragionamento possa essere fatto, per evitare che ci ritroviamo a litigare e creare dei conflitti sul 17 marzo, piuttosto che sul 4 novembre,

Vogliamo e dobbiamo discuterne per tempo, e secondo me dobbiamo rimettere a regime, nell'interesse generale del Paese, la problematica delle festività, con senso di responsabilità, anche perché essa sia utile

se quei fondi, che sono stati previsti e accantonati, erano in effetti ulteriori rispetto a quelli che poi sono stati resi pubblici attraverso notizie di stampa e che cosa avverrà

con l'auspicio di poter arrivare ad un consenso a 360 gradi per l'adozione di questo ordine del giorno, credo che in questo caso il problema si ponga.

«Il Senato della Repubblica, premesso che: un provvedimento per il riordino delle festività nazionali italiane appare necessario e dovrà essere basato sul rispetto delle tradizioni civili e religiose proprie delle ricorrenze nazionali, e includerà la celebrazione del 17 marzo, giornata dell'Unità d'Italia; non dovrà prevedere ulteriori giornate di vacanza scolastica né di astensione dal lavoro; d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dovrà inoltre consentire una più efficace programmazione delle vacanze scolastiche, oltre che dei periodi di ferie, al fine di sostenere l'industria turistica nazionale, anche attraverso una maggiore flessibilità delle ferie disposte nel corso dell'anno, al fine di incontrare la crescente domanda di brevi periodi dell'anno, al fine di incontrare la crescente domanda di brevi periodi di vacanza ed incentivarne lo svolgimento sull'intero territorio nazionale, impegna il Governo ad assicurare, per quanto di competenza, il proprio supporto ad ogni iniziativa, definita entro il 2011, anche di carattere legislativo, volta al riordino delle festività nazionali italiane».

dell'Istituto tecnico industriale statale «Luigi Trafelli» di Nettuno, in provincia di Roma, a cui diamo il benvenuto da parte del Senato.

si tratta di una norma tecnicamente necessaria e anzi va ringraziato il relatore, senatore Pastore, di essersi adoperato per trovare una formulazione che, senza creare problemi di copertura o di altro genere, sistemi i problemi che sarebbero emergere. Ricordo insieme a lui che già un anno fa si è provveduto, più che tempestivamente, con norma di legge, a prevedere

un clima di amarezza nel momento in cui gran parte del dibattito, relativamente all'adozione di questo provvedimento, si è incentrata

argomento. Composta la questione economica e quella amministrativa, sarebbe stato più giusto che la celebrazione e la solennizzazione di una giornata come questa si fossero rispecchiate in una norma asciutta, in cui le conseguenze di ordine amministrativo-organizzativo fossero state rimesse ad altro provvedimento di rango minore. Con tali sentimenti, che spero possano essere condivisi da buona parte dell'Assemblea, esprimeremo senz'altro su questo necessitato emendamento un voto favorevole.

anche le imprese a cui non si applica l'accordo interconfederale (che è fonte dell'obbligo retributivo nel settore privato) devono intendersi obbligate al pagamento della retribuzione per il 17 marzo. Prego, senatore Pastore.

un voto "anomalo" ma rispettabilissimo nella Commissione è stato approvato questo emendamento. Io ero contrario ed allora invitai al ritiro, perché ritenevo non vi fossero i presupposti di urgenza. Però intervengo anche nel merito, come ho detto prima, innanzitutto perché una festa dell'Unità d'Italia c'è già ed è quella del 4 novembre, che nel 2012 sarà automaticamente ricostituita senza bisogno di alcun intervento normativo; in secondo luogo, perché una giornata non festiva come tante ce ne sono porrebbe in secondo piano questo avvenimento così importante. Mi sembra quindi che contraddirebbe

credo di aver inteso che, essendo un emendamento votato in Commissione, il parere della Commissione è favorevole. Il relatore ha fatto delle considerazioni, che il Governo condivide, nell'illustrare i motivi del suo parere contrario. Il parere è contrario perché il provvedimento in esame tende a festeggiare 150 anni dalla creazione dello Stato unitario. L'Unità d'Italia è celebrata il 4 novembre; per quanto riguarda l'indipendenza - qui è il sardo che parla - noi indipendenti eravamo prima del 17 marzo 1861, e indipendenti anche dopo. Non confondiamo l'indipendenza con la creazione dello Stato unitario. Signora Presidente, mi rivolgo al collega Pastore, di cui da tempo apprezzo la correttezza e ovviamente anche la conoscenza dei Regolamenti e della prassi. Egli è relatore della Commissione come ha ricordato opportunamente il Sottosegretario, ahimè, il parere del relatore non può essere che favorevole rispetto ad un emendamento approvato dalla Commissione. La sua convinzione personale è nota e l'ha espressa ieri in Commissione, ma il parere del relatore in quanto relatore non può che essere ovviamente favorevole. I senatori del Partito Democratico voteranno a favore di questo emendamento nella considerazione che la giornata del 17 marzo, che ha registrato uno straordinario consenso nell'opinione pubblica del Paese, può continuare a vivere come un momento in cui ogni anno viene ricordato, soprattutto nel mondo scolastico, il valore della indipendenza del Paese - un valore alto, che animò il Risorgimento - e il valore della indivisibilità della Repubblica. Questo è il senso dell'emendamento che tende a far sì che, soprattutto nel mondo della scuola, il 17 marzo venga ricordato come un momento di riflessione sugli elementi fondanti della unità del Paese. *(Applausi

ma l'Italia ha iniziato ad affrancarsi dagli invasori stranieri e dallo Stato Pontificio con i primi moti insurrezionali all'inizio dell'800, e tutto è arrivato a conclusione dopo la Seconda guerra mondiale, nei confini che oggi conosciamo. L'indipendenza della Nazione non ha nessun motivo di essere ricordata in questo provvedimento, tantomeno l'insistenza sulla necessità della indivisibilità della Repubblica attraverso la proclamazione della Giornata nazionale. Quindi mi asterrò

onorevoli senatori, faccio seguito a quanto mi sono permesso di dire nella dichiarazione di voto sul primo emendamento, di tutt'altra portata naturalmente Non vi è alcuno, meno che meno da parte del nostro Gruppo, che possa essere contrario a sottolineare, valorizzare e celebrare l'indipendenza della nostra Nazione e del suo Stato sovrano e il valore dell'indivisibilità della Repubblica, dello Stato, della Nazione,

cercando di andare a speculare su presunte sensibilità diverse tra questo o quel Gruppo dello stesso schieramento sarebbe veramente di respiro corto e non renderebbe un buon servizio a questa giornata.

ma che spesso sono la sovrapposizione l'una all'altra di cose equipollenti o quasi identiche, di valori anche largamente condivisi ma che non si giovano della moltiplicazione e dell'ufficializzazione delle ricorrenze. finiscono, come prima giustamente il senatore Pastore ci ha ricordato, per inflazionare tali ricorrenze, per depotenziare e derubricare il valore di queste solennità,

è stato già ricordato, ci sono giornate solenni - in particolare il 4 novembre e il 2 giugno - già opportunamente accorpate al giorno festivo immediatamente successivo: sono delle date fortemente evocative del valore

non è unità meramente territoriale, non è solo confluenza di date, non è solo aggregazione di interessi, ma è comunità di destino, di provenienza e di desiderio di futuro, un destino scelto insieme e insieme perseguito e che legittima anche l'ordinamento statuale, l'ordinamento repubblicano, perché è comunità di civiltà e di storia. Quindi, ci sono già una quantità di ricorrenze che celebrano questi valori;

davvero la necessità di stabilire, ormai, nella nostra storia - non antichissima come comunità nazionale organizzata, ma tuttavia antichissima dal punto di vista della storia e della civiltà

Si mettono insieme, poi, l'indipendenza e l'indivisibilità, che sono valori diversi se la vogliamo dire tutta, e quindi anche dal punto dell'interpretazione e dei titoli si può dare luogo ad una qualche confusione. una qualche confusione. Noi dobbiamo volere, credo di poter dire, poche giornate, poche solennità adeguatamente enfatizzate, tali da coinvolgere realmente con una festività a tutti gli effetti, con giornate in cui non si stia a distinguere se sono lavorative o meno, perché quando una giornata è lavorativa si ha un bel fare appello alla celebrazione e al coinvolgimento della comunità nazionale: ognuno va al lavoro, ognuno privilegia la quotidianità delle sue incombenze. incombenze. E allora, poche festività. Ecco perché si è fatto già in precedenza uno sforzo di concentrazione sulle festività soppresse, sulle festività riunite. Poche, condivise, grandi celebrazioni... E questa è la quotidianità a cui infatti si dà la precedenza, è così. Le festività nazionali passano dopo, il treno parte e le altre incombenze incombono. È la riprova che sono giuste le osservazioni del relatore ed è giusto il parere contrario a questo emendamento. Signora Presidente, non tedierò a lungo l'Assemblea. Questo evento dimostra che il caso ogni tanto incombe anche su quest'Aula. La Commissione ha votato questo emendamento e, secondo me, ha fatto bene a votarlo. E votandolo, in un certo senso, ha tolto forza alle obiezioni che i colleghi oggi ci presentano,

a cui vogliono invitarci i colleghi della maggioranza, non tenga conto proprio di questo. Il Parlamento dovrebbe essere in sintonia con ciò che accade nella soggettività sociale; si è visto e si è toccato con mano come la soggettività sociale abbia riscoperto, a distanza di molti anni, collettivamente, con una sorta di allegrezza imprevista,

rapidamente attirare l'attenzione sul concetto della indivisibilità. Il mio timore è che gli oratori

indivisibilità abbia un significato pregnante e costruttivo, che si pone in modo alternativo a una visione distorta del federalismo. Il federalismo è altro,

L'articolo 5 della Costituzione così recita: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali». Questa, peraltro, è la lezione del presidente Napolitano.

avviso, il 17 marzo non può essere considerata la Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione e della Indivisibilità della Repubblica.

testuali. Quindi io credo che fin da allora ci sia stato un atteggiamento molto diverso, e che l'unità della Repubblica, così come ha già detto il senatore Rutelli, vada festeggiata il 2 giugno. Che poi recuperare nelle scuole, nella società, il valore dell'insediamento del primo Parlamento nazionale - primo Parlamento italiano sia un compito della società civile, delle istituzioni, delle scuole (perché no?), che dovrebbero insistere molto di più sull'insegnamento della storia, sia un dovere nazionale, non riconducibile alla retorica che qui in Parlamento ci ha sfinito, è

a pochi minuti o a depositare i propri interventi scritti sarà possibile procedere al voto finale per le ore 13, diversamente occorrerà rinviare la votazione ad un'altra seduta.

anche l'Unione di Centro è d'accordo sul rinvio delle

spesso in quest'Aula vengono citate alcune istituzioni, come la Banca d'Italia, quale modello di serietà, prestigio ed autorevolezza; al contrario, quanto avviene al loro interno è una situazione da sepolcro imbiancato, dove l'opacità e l'impermeabilità rappresentano la regola, anche nella gestione dei concorsi interni, accusati da alcuni sindacati di possibili brogli. In un comunicato sindacale intitolato «Le Giunte dei Rabdomanti», infatti, il Sindacato indipendente della Banca centrale ha avanzato critiche e dubbi sul funzionamento delle giunte di scrutinio delle carriere direttive in merito a concorsi interni manipolabili. «Con quali criteri sceglie la giunta?», chiede il sindacato, rimarcando che, salvo che Bankitalia non abbia dotato i commissari di appositi bastoni da rabdomante, mancano i presupposti per verificare le attività delle giunte di scrutinio. Da documenti acquisiti, e tradotti in un'interrogazione parlamentare, la 4-04822, signora Presidente, colleghi, risulta che alcune commissioni avrebbero inviato le tracce dei temi ad alcune persone, tra cui il responsabile della vigilanza della sede di Brescia, dottor Cannistraro, nominato nella commissione nel 2007 dal capo della vigilanza, dottoressa Anna Maria Tarantola, proprio fiduciario sulla piazza

sarebbero circolate tracce di temi ed informazioni riservate sulle prove, ad esclusivo appannaggio di raccomandati, penalizzando i candidati più preparati e più meritevoli, Continuerò, signora Presidente, a denunciare opacità ed illegalità diffuse all'interno di Bankitalia e le malefatte di una gestione molto poco trasparente da parte di una cricca di potere che va a braccetto con i banchieri,

ai rappresentanti eletti dal popolo, che vogliano chiedere trasparenza; e il signor governatore Draghi all'interno continua a far fare tutto quello

settimana scorsa i Comuni di Soave e di Monteforte d'Alpone, dopo la gravissima alluvione del novembre scorso, si sono trovati di nuovo in una condizione sconfortante; le assicuro che non ho alcuna voglia di

davvero chiediamo al Governo di supportare la Regione Veneto, se non basta il commissario da solo. Mi rendo conto che un commissario può adottare procedure che nella transizione e nell'emergenza non esigano i tempi lunghi dei progetti sostanziali, strutturali e di lungo termine: ma almeno i canali scolmatori! Almeno un aiuto! Usiamo i militari per tutto, in Italia, anche per fare

che lo vede operare con un *team* di tecnici assolutamente qualificati. Sono quindi convinto che la Regione Veneto abbia la capacità e le potenzialità di intervenire per far fronte a queste necessità.